Signora Presidente, non chiederemo la verifica del numero legale,

Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 20 luglio 2017 Onorevole Presidente, informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Enrico COSTA dalla carica di Ministro senza portafoglio. *F.to* Paolo GENTILONI».

Signora Presidente, la mozione che abbiamo presentato per primi in questa sessione di attività dei lavori del Senato riguarda la tutela del riso prodotto in Italia.

di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea. La produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa,

Nel 2026 tali importazioni arriveranno, se non ci si ferma, a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Con questi ritmi si produce un semplice effetto: chiudono i produttori italiani.

deformazioni all'interno del mercato tali da produrre - come ho già anticipato - la chiusura, la perdita di quote e di produzione all'interno del mercato europeo. Il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi, con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per giungere all'imposizione dei cosiddetti dazi. L'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi effetti negativi molto gravi nei confronti della nostra produzione, che si concretizzano nella marcata riduzione delle superfici coltivate a riso. Signora Presidente, in estrema sintesi, con la mozione n. 746 chiediamo al Governo, anche alla luce degli ultimi sviluppi,

per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA; 2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente; 3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e

in questo caso, fanno *dumping* nei confronti dei nostri produttori di riso. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il settore risicolo continua a essere oggetto di attenzione del Parlamento. Risale al luglio del 2014, infatti, un importante lavoro della 9a Commissione del Senato che ha portato all'approvazione di una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del comparto risicolo italiano. Nel corso degli ultimi anni diverse sono state le interrogazioni relative alla crisi del settore del riso. Il legislatore ha assunto un atteggiamento propositivo predisponendo una delega per riformare la normativa nazionale del settore (risalente al 1958), che è stata inserita nel cosiddetto collegato agricolo, sulla base della quale, proprio in questi giorni, il Governo ha emanato il relativo decreto legislativo, tenendo conto dei contenuti e anche del prezioso giudizio positivo di buona parte della filiera audita e ottenendo il parere favorevole delle Commissioni competenti. Il nostro Paese - come si è detto - è il principale produttore europeo di riso, con un fatturato annuo di un miliardo di euro, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere ad alta specializzazione. Le peculiarità della filiera risicola europea le permettono di differenziarsi da quelle del resto del mondo. L'elevata specializzazione di alcune imprese di settore conferisce al comparto risicolo europeo un importante ruolo di gestione delle acque, garantendone disponibilità a lungo termine. Gli operatori del comparto, inoltre, sono molto attenti alla salvaguardia dell'ambiente e, attraverso il loro lavoro, contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali,

L'impegno del Governo è stato conseguente e ha portato a predisporre un *dossier* presso la Commissione dell'Unione europea che descrive le problematiche del settore. È seguito, poi, lo scorso febbraio, un importante incontro tra tutti i Paesi produttori di riso, grazie a un'iniziativa presa dal nostro Paese, che ha avuto lo scopo di raggruppare e rafforzare il ruolo e la posizione dei produttori interessati, con il coinvolgimento delle autorità politiche e dei rappresentanti degli operatori di tutta la filiera dell'Unione, e ha dato vita all'istituzione della European rice platform, ove è stata condivisa la necessità di rendere quanto più trasparente possibile l'intero processo di produzione che riguarda il riso italiano, sperimentando l'indicazione dell'origine in etichetta. Su questo punto, l'intervento del Governo, teso ad anticipare le decisioni della Commissione europea - ancora prende tempo sull'attuazione della normativa in materia di etichette trasparenti - con il decreto sull'etichettatura del riso della settimana scorsa dà conto (rispetto anche ai contenuti della mozione) della piena condivisione delle linee d'indirizzo che, nel corso del tempo, sono maturate all'interno della maggioranza. E per questo un ringraziamento al Vice Ministro, che è qui presente, e al Governo. L'Italia ha deciso di intervenire per garantire massima trasparenza in etichetta sulla provenienza del riso. Dalla scorsa settimana, infatti, l'indicazione del Paese d'origine in etichetta diventa obbligatoria anche per la pasta e il riso, dopo le norme analoghe in materia di latte e formaggi. Sarà una sperimentazione che durerà due anni, nel corso dei quali il nostro Paese sarà comunque chiamato a impegnarsi affinché questa volta sia la normativa europea a equipararsi a quella italiana. Dobbiamo essere fieri del coraggio che la maggioranza di questo Parlamento ha avuto nell'affrontare con forza e determinazione il problema

quella del riso è una filiera composta da più di 4.200 aziende, che si occupano di coltivazione e si trovano perlopiù nella parte settentrionale dell'Italia, con un'alta concentrazione in Piemonte e Lombardia. un comparto che conta anche numerose industrie di lavorazione e che in totale vanta un giro di affari di circa un miliardo di euro. In tutto questo va sottolineato che su scala europea l'Italia riveste un importantissimo primato: il nostro Paese è il primo produttore di riso, con un territorio investito in questa coltivazione pari a 237.000 ettari. Lo stivale tra l'altro rappresenta un vero e proprio esempio a livello mondiale, perché ha creato e migliorato la varietà originale, in modo da adattarla al territorio e alle tradizioni locali. Nonostante questo, però, il settore risicolo nazionale sta vivendo una crisi assai seria, che si è aggravata nel corso degli ultimi anni a causa dell'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, coadiuvato dal sistema di preferenze generalizzate. Questo sistema, nato per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, ha però di fatto cagionato la riduzione dei prezzi di mercato del riso prodotto in Italia e all'interno dell'Unione europea al di sotto degli stessi costi di produzione, determinando forti danni alle imprese italiane; una crisi certificata dalla Commissione europea, che ha preventivato per la campagna in corso rimanenze finali (cioè di prodotto non collocato sul mercato) pari a 585.000 tonnellate, vale a dire circa un terzo dell'intera produzione comunitaria. La risicoltura italiana rischia dunque di essere fortemente ridimensionata, mettendo in serio pericolo un vasto territorio e tutta la connessa filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche e occupazionali, ma anche ambientali e sanitarie. Nello specifico, le ricadute ambientali si collegano alla compromissione dell'ecosistema e dell'equilibrio idrogeologico, proprio per via dell'abbandono dei terreni coltivati. Le conseguenze sanitarie, invece, si legano al fatto che in tantissimi prodotti di origine asiatica è stata più volte rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati, e ciò espone i consumatori a inevitabili rischi che pregiudicano irreversibilmente la sicurezza alimentare. Ora, sotto il profilo strettamente nazionale, va precisato che le varietà di riso italiane possiedono specifiche proprietà, legate ai luoghi e alle tecniche con cui avviene la coltivazione. In questo senso, preservarne e difenderne l'esistenza è importante per custodire una lunga tradizione agricola, per potenziare le caratteristiche legate alla trasformazione della lavorazione in cucina del prodotto e per conservarne la tipicità gastronomica. Si tratta di una peculiarità che è importante ricordare ed è uno dei sintomi delle eccellenze italiane nel mondo. È evidente che il valore della filiera risicola italiana risiede proprio nella strategicità territoriale e nella protezione della preziosa biodiversità del prodotto. Questo contribuisce a mantenere alta l'immagine del *made in Italy* alimentare, assicurando la stabilità socioeconomica di un complesso territoriale di assoluta

informazioni concrete, chiare e non fraintendibili sui requisiti, sulle caratteristiche e sulla qualità del bene alimentare che sta acquistando e che sceglie di mangiare. Il riso, prima ancora di essere una vera e propria ricchezza dal punto di vista agricolo, rappresenta un patrimonio culturale, parte fondante delle nostre tradizioni e della nostra identità. Non ci stancheremo mai di ricordarlo e continueremo ovviamente a lottare senza sosta contro ogni tipo di svendita delle nostre inestimabili risorse

Il tema del caporalato rimane tuttora, nonostante la legge che abbiamo approvato, molto attenzionato;

2015, a seguito di un'intensa attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro - Commissione che presiedo - dell'indagine aperta sulla morte della signora Paola Clemente, nonché di un sopralluogo-ispezione compiuto nella zona dell'Agro Pontino il 24 maggio forestali, impegna il Governo: 1) a rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri. Come dicevo prima, anche i controlli e gli arresti avvenuti questa mattina vanno in siffatta direzione. Il secondo impegno è volto a operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo. Per quanto contenuto nella normativa, possiamo dire che ancora non vi è una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro in coordinamento con le ASL. Abbiamo inserito nella mozione anche l'impegno a effettuare la vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli

possibilità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione

dei lavoratori agricoli, che la sorveglianza sanitaria è sostituita da una certificazione medica preventiva valida per due anni e che la formazione in materia agricola è sostituita dalla mera consegna di documenti. Concludo l'illustrazione delle presente mozione dicendo che, nel caso specifico,

oggettivamente, sul piano della salute, è molto complicata.

signori del Governo, colleghe e colleghi, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, lo scorso mese di novembre

il perimetro dentro il quale ci si deve muovere all'interno delle organizzazioni dell'imprenditoria agricola, con livelli di chiarezza che possano ancora di più e in modo migliore rappresentare un'efficace condizione di contrasto alle attività illecite e allo sfruttamento del lavoro. Ricordo che l'*iter* parlamentare di questa legge si è svolto in un clima di grande partecipazione, ma anche di grande emozione, determinata proprio dalla morte

del lavoro in agricoltura e sull'azione di repressione che si consegue attraverso la riscrittura dell'articolo 603-*bis* del codice penale, con la previsione della confisca dei beni e dell'arresto in flagranza di reato. Invero, nella legge è precisato che le condizioni afflittive più pesanti che sono state introdotte ricorrono soltanto in presenza di due condizioni, e cioè lo sfruttamento del lavoratore e l'abuso dello stato di bisogno del lavoratore La sanzione penale parrebbe, di conseguenza, non applicabile nei casi in cui vi sono violazioni accidentali, ovvero infrazioni correlate a lievi inadempienze. pare che così non sia e c'è uno stato di particolare ‑ e io ritengo anche motivato ‑ preoccupazione da parte di tutto il mondo agricolo. Mi permetto di ricordare che opera nel nostro Paese circa un milione di imprese agricole: nella mia Puglia sono 80.000; nel Mezzogiorno d'Italia sono 330.000. L'agricoltura nel nostro Paese pesa il 2,2 per cento del PIL; 12 milioni di ettari sono utilizzati in agricoltura e gli occupati raggiungono presenze, rappresentando il terzo valore più alto nell'Unione europea dopo la Polonia e la Romania. questo per evidenziare come e quanto il comparto agricolo rappresenti un motore di sviluppo dell'occupazione e di sostegno al PIL, il che - evidentemente - impone di fare chiarezza su alcuni punti, che possono rappresentare

sugli argomenti inerenti il comparto agricolo. Abbiamo parlato della necessità degli snellimenti dei processi e, quindi, della minore burocrazia, della semplificazione delle procedure, della necessità della tracciabilità delle produzioni,

all'uso delle risorse del Fondo anti-tratta anche per i reati di cui al medesimo articolo, si è inserito nel nostro ordinamento, per la prima volta, il reato di sfruttamento lavorativo, riconoscendo una responsabilità specifica anche alle imprese e non soltanto a chi esercita l'intermediazione illegale di manodopera. sfruttamento del lavoratore, ossia l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Molti problemi sono stati sollevati in relazione alla questione degli indici di sfruttamento, confondendoli come elementi costitutivi del reato. Non è così, in quanto gli indici erano presenti anche nella vecchia scrittura dell'articolo Il ricorrere di singole violazioni non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Anzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, essi costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento, che implica, invece, una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati e tutelati.

che necessariamente si sviluppa nel tempo e integra una situazione di fatto duratura e non contingente. È del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento «ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro» (sto citando da una serie di interventi). Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei a inibire o limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'approfittamento, l'approfittamento, appunto, dello stato di bisogno in cui versa; uno stato che, per definizione, esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale. Il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione - sto parlando dell'articolo 36, 1, della Costituzione - limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3 della Costituzione), diritto alla sicurezza sul lavoro e alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana. Per quanto riguarda la parte penale, bisognerà sicuramente monitorare l'andamento della legge per verificare eventuali problemi e necessità di aggiustamento. Invece, nella parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, registriamo un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano le linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni. Inoltre, in alcune zone del Paese registriamo ancora la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate sia nella raccolta stagionale dei prodotti agricoli sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni. Ricordo soltanto gli ultimi episodi gravi di Rosarno e San Ferdinando, dove ci sono stati morti, e i casi, comunque gravi, registrati in Toscana, nel Chianti, in Emilia Romagna e in Provincia di Forlì-Cesena. È in questo quadro che chiediamo al Governo se non ritenga di fare il punto della situazione e di impegnarsi a costruire gli strumenti necessari affinché anche la parte preventiva della legge, legge, in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze e indirizzare le scelte di intervento future, venga attuata completamente. Inoltre, bisogna ipotizzare un piano di intervento che preveda misure per l'accoglienza, la sistemazione logistica e il supporto ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti locali e delle associazioni. Il punto è che con le sezioni territoriali, che vanno organizzate, della rete per il lavoro agricolo di qualità,

Signora Presidente, lo scorso 18 ottobre 2016 veniva approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge n. 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», diventato la legge n. 199 del 29 ottobre 2016. Con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. Le principali novità della legge riguardano la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. Legge a parte, è evidente che il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili per uscire, una volta per tutte, dalla '"ghetto *economy*". Infatti, la legge n. 199 del 2016 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo resta soprattutto da colmare il *gap* di un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra la domanda e l'offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato; ad oggi, infatti, sono ancora inattuate alcune misure specifiche previste dalla legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura e sono tanti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, tutte questioni che vanno risolte, perché si tratta di un sistema che non è più tollerabile, sotto tutti i punti di vista. Farsi trovare nuovamente impreparati davanti a una raccolta estiva già iniziata significherebbe sferrare l'ennesimo colpo alla dignità dei lavoratori stagionali e non possiamo assolutamente permetterlo. *(Applausi

Anche il mondo dell'edilizia e alcuni comparti dei servizi vivono la stessa drammatica esperienza del caporalato. La legge n. 199 del 2016 interviene allargando la fattispecie penale, ma non generalizzando.

indiscriminato, di fronte a semplici e futili divergenze, inadempienze o irregolarità. richiede che vi siano due elementi, entrambi necessari, per configurare il reato di caporalato: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittarsi dello stato di bisogno. È stata anche corretta da parte di diversi colleghi - segnalo in modo particolare l'intervento della senatrice Gatti - l'interpretazione secondo cui gli indici non sarebbero elementi costitutivi del reato. Si deve trattare di una reiterazione delle condotte e delle violazioni e gli indici sono semplicemente degli indicatori che

Signora Presidente, cinque minuti sono pochi per riuscire a riassumere un tema impegnativo e importante come la necessità di tutelare la filiera del riso.

In tal senso l'Italia non deve fare solamente all'ultimo istante i compiti a casa, ma deve far valere le proprie ragioni fin dal primo momento. La difficoltà che sta vivendo il nostro settore

a più riprese e l'ultima volta qualche mese fa, ha scritto che già da diversi anni l'Ente nazionale risi sta chiedendo alla Commissione europea di applicare la clausola di salvaguardia, che nella regolamentazione attuale ha lo scopo di ripristinare i normali dazi di importazione; e non perché dobbiamo essere cattivi nei confronti dei Paesi meno avanzati, ma perché è evidente che lo svantaggio che stiamo subendo è solo italiano e non di altri Paesi europei. La collaborazione e la partecipazione dell'Unione europea nei confronti dello sviluppo economico di tali Paesi corrisponde a un prezzo pagato dall'agricoltura italiana,

ha iniziato a farsi vedere presente e a far capire che qualcosa forse va fatto. La cosa ci ha molto deluso, perché abbiamo seguito la questione nei mesi passati. E, quando

in sede europea a trattare e difendere il settore risicolo, ma - come purtroppo abbiamo visto e appreso dai documenti - a Bergamo, per sostenere la propria candidatura e il proprio *ticket* con Renzi,

il ministro Martina era assente ingiustificato. Queste cose ci fanno male

non solo lo sfruttamento del lavoratore, ma anche il fatto che esso sia ottenuto attraverso l'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore stesso: si assegna cioè importanza alla situazione di vulnerabilità della persona vittima di sfruttamento.

è particolarmente forte - e da associazioni di volontariato, che pure si occupano di siffatti temi - la Caritas, Proxima e altre - apprendiamo che in varie zone d'Italia, in agricoltura, il lavoro femminile è sottoposto a un regime di sfruttamento e di ricatto particolarmente feroce. Ciò dipende proprio dalla maggiore debolezza delle donne nel rapporto di lavoro

quindi giusto presidiare al massimo questi temi. rapporto di lavoro è legata anche al sovraccarico di lavoro domestico e di cura e alle condizioni disumane in cui sono costrette a lavorare, senza sostegno pubblico - ad esempio per la cura dei figli - e ad altri fattori connessi al tipo di lavoro che svolgono. Mi riferisco in particolare al fatto che i braccianti,

si realizza una spinta alla prostituzione coatta, soprattutto delle giovani donne immigratem che sono deboli sotto due profili: perché donne e perché immigrate. Abbiamo dati drammatici noti che riguardano Ragusa, ma anche altri posti, dove si registra un tasso di aborti

Tra le eccellenze da tutelare vi è senza dubbio la coltivazione del riso, che nel nostro Paese è indissolubilmente associato alle più ricche e storiche tradizioni regionali, in particolare culinarie. Indubbiamente, le caratteristiche del riso prodotto in Italia rispondono a parametri qualitativi che non sono rintracciabili altrove nel mondo. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed il relativo comparto ha plasmato intere aree della nostra penisola, garantendo anche un buon bacino di occupati. La valorizzazione della produzione risicola italiana significa da una parte tutelare tali elevati standard qualitativi, dall'altra non abbandonare i territori produttivi e i consumatori italiani. Pertanto sarebbe necessario attivarsi con più energia in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente, oltre ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "*made in Italy*".

sottopagati e senza tutele: bisogna adoperarsi affinché si rafforzino i controlli interforze e si garantiscano forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività i lavoratori stranieri; inoltre, un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL ed un potere di sorveglianza più idoneo sulle agenzie di somministrazione sarebbe auspicabile per una vigilanza efficace in materia di sicurezza del lavoro agricolo. Abbiamo già cercato, in questa legislatura, di contrastare il fenomeno del caporalato. Ora dobbiamo continuare ad adoperarci per il completamento della cabina di regia nazionale, e per la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori. Lo sviluppo del settore agricolo non può prescindere da queste azioni e aspetti. Per concludere, stiamo positivamente mettendo in campo un modello di agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione, stiamo delineando nuove traiettorie di futuro per un comparto fondamentale per l'economia nazionale ed europea, al fine di tutelare l'ambiente e gli equilibri idrogeologici e di salvaguardare la ricchezza della nostra biodiversità vegetale e animale. Questa è una fase storica cruciale per aumentare la velocità di questi processi virtuosi e fare del nostro Paese l'esempio in Europa e nel mondo di potenza agricola responsabile. Non possiamo fermarci proprio ora e pertanto auspico un'azione risoluta del Governo in tale ambito.

e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente che rispetti i diritti sociali, i diritti dei lavoratori e tuteli l'ambiente. Nell'ambito della prossima

Deve essere promossa la conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai affermate e stimate sui mercati mondiali, soprattutto per i suoi virtuosi

È altresì importante l'avvio, con le risorse che si renderanno disponibili, di campagne promozionali per incrementare il consumo di riso italiano nell'Unione europea, un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra economia agricola e a cui va dato il giusto risalto. È poi necessaria la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, prima tra tutti la pubblicità ingannevole e quella comparativa illecita,

Vanno poi adottate iniziative che prevedano l'estensione dell'assicurazione sui ricavi del grano anche alla filiera del riso italiano, per costituire finalmente una rete protettiva che assicuri il reddito degli agricoltori. Occorre promuovere iniziative tese a valorizzare il riso italiano prodotto e lavorato direttamente dagli agricoltori (oppure, in delega a lavoratori terzi). Il nostro riso, dunque, deve essere immesso nel mercato locale tramite una filiera diretta ed una vendita in sede attraverso agriturismi (o equiparabili), oppure nei circuiti di vendita associativi, in modo da preservare l'identità e la tipicità della filiera locale tra produttore e prodotto. È infine necessario adottare tutte le azioni utili a non disperdere la particolare tradizione della coltura risicola italiana; il tutto, ovviamente, nell'ottica di una semplificazione del sistema di etichettatura dei prodotti che deve sempre - lo ripeto puntare alla massima chiarezza e trasparenza. Si tratta di azioni imprescindibili che devono essere adottate in tempi rapidi, affinché il comparto risicolo italiano possa essere concretamente tutelato. Concludo con lo slogan dell'anno internazionale del riso, una celebrazione che si è svolta per l'intero 2004, secondo il quale: «Il riso è vita». questo motto tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno tentato di massacrare il comparto risicolo italiano; un comparto che deve essere sottratto alla concorrenza selvaggia di affaristi senza scrupoli scrupoli e che rappresenta davvero vita e sostentamento per tantissime persone che operano nel settore, che merita di essere sorretto e supportato con grande forza,

che ho sottoscritto con altri colleghi, impegna il Governo a vigilare sulla concreta attuazione della legge di contrasto a fenomeni di caporalato in agricoltura; un fenomeno dalle ampie e preoccupanti dimensioni che comporta condizioni di sfruttamento dei lavoratori incompatibili con i diritti fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale; un fenomeno strutturato e organizzato. Il caporalato in agricoltura, ma anche in altri settori, costituisce violazione alla Costituzione italiana e ai fondamentali diritti del lavoratore: è sfruttamento, perché perché il lavoratore non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e perché comunque non dispone di una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata della giornata lavorativa supera di norma quella stabilita per legge e il lavoratore non gode del riposo settimanale e di ferie retribuite, come sancito dai commi secondo e terzo dell'articolo 36 della Costituzione. Non parliamo poi del mancato rispetto dei limiti di età e delle mancate tutele per le lavoratrici madri, Le premesse che ho poc'anzi enunciato sono correlate all'impianto della legge n. 199 del 2016, che comporta modifiche al codice penale; in particolare, faccio riferimento all'articolo

lavoro con modalità di sfruttamento, violenza o minaccia. Tale formulazione si era dimostrata, nel corso dei cinque anni trascorsi precedentemente alla presente legge, del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno. scaturita la necessità di introdurre modifiche all'articolo 603-*bis*, con la riscrittura della condotta dell'intermediario e la punizione anche del datore

la previsione del reato autonomo del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo, anche senza il ricorso a un intermediario. Degno di nota è il fatto che la legge introduca nel codice penale l'ipotesi di circostanze attenuanti specifiche per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, premiando forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che aiutino ad estirpare il fenomeno Inoltre, il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, previsto dalla legge n. 199, diviene un importante strumento di controllo e di prevenzione del lavoro irregolare in agricoltura, in particolare per i lavoratori stranieri con lavori stagionali. Fondamentale è dunque il funzionamento della rete con una struttura articolata sul territorio, attraverso nodi locali o sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti in convenzione. Con tale ampia struttura partecipata sarà disponibile la conoscenza di dati sulla quantità, capacità, qualità e specializzazione della manodopera disponibile alle esigenze del territorio e alle caratteristiche delle produzioni, al fine dell'ammodernamento dei sistemi produttivi. Il piano di attuazione della legge prevede inoltre il coinvolgimento delle amministrazioni statali, Regioni, Province autonome, amministrazioni locali e terzo settore. Tale cooperazione è e deve essere accompagnata da azioni di monitoraggio dell'efficacia dei provvedimenti attuati per combattere questo fenomeno strutturato. Ben venga dunque l'impegno chiesto al Governo di verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, la cui forza dissuasiva necessita sì di tempi lunghi per apprezzarne i benefici, ma in tempi brevi deve trovare le modalità più congrue per sostenere dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli, nonché forme sperimentali per attivare nodi

Naturalmente, nel formulare i pareri, mi riferirò in particolare agli impegni contenuti nelle diverse mozioni più che all'insieme del dispositivo in premessa.

«ad effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;». la seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;».

prima di procedere

l'elaborazione di linee guida per tutto il territorio nazionale, dirette agli organi amministrativi, che svolgono funzioni di accertamento nei settori interessati dai fenomeni di cui si tratta;».

a condizione che il punto 7) degli impegni venga riformulato come segue: «ad eseguire un monitoraggio volto a evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della nuova normativa e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere».

e comunque sullo stato d'attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno, con conseguente informativa alle Camere;». PRESIDENTE.

nella rete pubblica e privata dei servizi per il lavoro, con il coordinamento delle Regioni e sotto la supervisione di ANPAL;». Sul punto 11)

tra i requisiti ostativi o limitativi per accedere a risorse europee nel contesto della formulazione degli avvisi, bandi o graduatorie pubbliche, in linea con quanto previsto anche in altri settori dell'ordinamento».

si ripete nelle diverse riformulazioni.